L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, avverto che la prevista informativa del Governo sui gravi fatti della clinica "Santa Rita" di Milano avverrà domani mattina alle ore 11,30, con l'intervento del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, professor Ferruccio Fazio. I Gruppi potranno successivamente intervenire per cinque minuti ciascuno. Comunico che la 14a Commissione permanente ha proceduto in data odierna alla propria costituzione. Sono risultati eletti: Presidente: Boldi; Vicepresidenti: Santini e Pedica; Segretari: Sibilia e Di Giovan Paolo.

la costituzione delle Commissioni bicamerali - della cui composizione è stato dato annuncio nella seduta pomeridiana del 4 giugno scorso - avrà luogo giovedì 19 giugno prossimo nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario.

ore 13,30: Commissione parlamentare per le questioni regionali; Commissione parlamentare per l'infanzia; Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. ore 14,30: Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione; Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Onorevoli colleghi, sono trascorsi venti anni da quando, l'11 giugno 1988, veniva a mancare Giuseppe Saragat, quinto Presidente della Repubblica italiana, già Presidente dell'Assemblea costituente, padre nobile della socialdemocrazia italiana. Nato il 19 settembre 1898 a Torino, Saragat rappresenta una personalità di straordinaria vitalità intellettuale, capace di dirigere e guidare un partito, fino quasi a immedesimarsi completamente in esso, trasformarne le strutture portanti e determinarne le linee guida in un tempo lungo e difficile. La genesi e la storia del Partito socialdemocratico affondano le radici nel suo inesausto tentativo di riunificare le correnti del socialismo italiano prima e durante l'esilio che segue i primi anni di militanza nel Partito socialista unitario di Turati e Matteotti, cui si iscrive nel 1922, appena dopo la scissione di ottobre, accedendo alla direzione del partito, a soli 27 anni, nel 1925. La sua formazione culturale - lo ricordava il presidente Spadolini nella commemorazione tenuta in Senato il 14 giugno del 1988 - si fonda su influenze nobili e composite: Turati e Treves, Croce ed Einaudi. La decisiva esperienza dell'espatrio tra il 1926 e il 1943 e poi della Resistenza contribuisce allo sviluppo del suo modo di intendere il socialismo in chiave umanitaria e riformista riformista intransigente, si vorrebbe dire - e lascerà segni durevoli nella sua concezione dell'Europa, delle fasi storiche dello sviluppo del continente, ma anche in una visione politica al tempo stesso equilibrata ed idealista, riassumibile nella frase per cui «non si può e non si deve rinunciare alla soluzione di un problema, solo perché questo ne pone altri parimenti difficili (...) ogni età e fase della storia pongono problemi solubili per il fatto stesso che la coscienza degli uomini li ha creati e fatti propri. Il rientro in Italia, cui seguono i mesi concitati dell'arresto, l'evasione e poi l'attivismo politico clandestino nel Partito socialista italiano di unità proletaria, costituisce il preludio di quella straordinaria carriera politica vissuta ed intesa sempre come proiezione costruttiva nella vita delle istituzioni democratiche. Percorso ricco, attraversato da suggestioni variegate e da un intarsio di esperienze che lo vedono prima ministro senza portafoglio nel II Governo Bonomi, nel 1944, poi anche ambasciatore d'Italia a Parigi, l'anno successivo. Il 26 giugno del 1946 è eletto Presidente dell'Assemblea costituente e conduce in modo esemplare tutta la prima fase della legislatura costituente, quella comunemente ribattezzata dell'unità nazionale, che contribuirà in modo determinante a gettare il seme fertile per il compimento dell'opera di redazione della Carta costituzionale. In qualità di Presidente, Giuseppe Saragat svolge un delicato delicato e paziente ruolo di mediazione tra le varie anime già emerse in seno alla Commissione dei Settantacinque, poi condotte ad ammirevole concordia e sinergia nell'ultima parte dei lavori dell'Assemblea, sotto la guida di Umberto Terracini. Nel pieno di quell'esperienza ricca, stimolante, sempre votata alla composizione dei dissensi in una prospettiva di fruttuosa collaborazione, pur nel riconoscimento delle reciproche differenze, anche nello stesso campo socialista, Giuseppe Saragat si trova di fronte ad un momento cruciale della storia politica del Paese, quando si rompe l'accordo tra la Democrazia cristiana ed i Partiti socialista e comunista. La sua contrarietà alla convergenza tra il Partito comunista ed il Partito socialista lo conduce, il 6 febbraio 1947, alle dimissioni da Presidente dell'Assemblea Costituente e alla scissione socialdemocratica di palazzo Barberini, che chiude definitivamente la fase dell'unità nazionale e prelude alla nascita di un nuovo soggetto politico: il Partito socialista dei lavoratori italiani. È questo uno snodo cruciale, in cui si intravedono i paradigmi di una sensibilità altissima, completata dalla piena consapevolezza di un'azione capace di conciliare i diversi livelli della vita del Paese, la strategia politica lungimirante, la salvaguardia e la salute delle istituzioni repubblicane proprio nel momento della nascita e poi del loro delicato e progressivo consolidamento. Infine, e soprattutto, la forza delle idee e la tenacia di quella dottrina socialdemocratica, europeista, umanitaria, liberale, atlantista che costituirà una delle matrici nobili che innerveranno di sé più di quattro decenni della vita culturale e politica del Paese. Sono queste le suggestioni che conducono Giuseppe Saragat alla fondazione, nel 1951, del Partito socialdemocratico italiano, del quale sarà guida risoluta attraverso le perigliose acque delle diverse fasi del centrismo prima e del centrosinistra poi. Egli sa farsi equilibrato interprete e protagonista di una posizione progressista e riformista nel panorama delle forze politiche nazionali, costruendo per il Partito socialdemocratico il ruolo di potenziale baricentro per un quindicennio, dal 1950 al 1964. Ed il peso del partito di Saragat è invero decisivo durante la ricostruzione centrista, in forza del suo fecondo rapporto dialettico con Alcide De Gasperi e poi, nella fase successiva, con Aldo Moro. Le nomine a ministro nei Governi degli anni Cinquanta e poi, via via, negli anni del centrosinistra segnano il progredire di un *cursus honorum* da cui origina il suo settennato da Capo dello Stato, che si apre con l'elezione avvenuta nel 1964, al ventunesimo scrutinio, e si chiuderà nel 1971. La straordinaria attualità della figura politica di Giuseppe Saragat vive nella visione dell'Europa, illustrata nel discorso di insediamento avanti al Parlamento in seduta comune, in cui egli ha ad affermare che «la costruzione di un'Europa democratica, economicamente e politicamente integrata, è un potente fattore di pace». E ancora, è doveroso soffermarsi sull'afflato straordinario con cui Saragat guarda alla Carta costituzionale democratica e pluralista - che con coraggio aveva contribuito a far nascere - quando ricorda, in un momento così delicato e complesso dell'attuazione dei suoi istituti «che non vi è priorità nella realizzazione dei dettati della Costituzione, tutti da attuarsi in armonico sviluppo, in rapporto ai mezzi disponibili». Il ruolo del Capo dello Stato, custode della Costituzione, si colora con Giuseppe Saragat di quel tratto di umanesimo che lo rende - sono le sue stesse parole nel messaggio agli italiani del dicembre del 1964 - «Presidente al di sopra dei partiti e un sereno moderatore dei contrasti che la vita del Paese sprigiona nel suo sviluppo». Con il 1971 ha termine un settennato in cui egli ha interpretato in modo rigoroso e sensibile il ruolo della più alta magistratura della Repubblica. Siede quindi in questa Assemblea come senatore di diritto e a vita in modo esemplare, declinando sempre la forza dei propri valori patria, libertà, umanità - anche nei momenti più oscuri e difficili vissuti dalle istituzioni repubblicane, attaccate dal terrorismo, dalla violenza, da - e sono ancora parole di Giovanni Spadolini - «i mostri e i deliri» del secolo scorso. La sua acclamazione a presidente del Partito socialdemocratico italiano, il 29 luglio del 1975, rappresenta, insieme con il ritorno all'impegno politico attivo, il mirabile coronamento di una vita costantemente percorsa da coerenza ed alta idealità e da una spiccata capacità di leggere con passione i complessi sommovimenti della società italiana e le dinamiche del mondo dei lavoratori. Onorevoli colleghi, certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, nel rivolgere un pensiero deferente alla figura di Giuseppe Saragat, ricordo le parole pronunziate nel 1925 da lui giovane; esse valgono forse oggi ancor più di allora: «La libertà è la premessa indispensabile di qualsiasi lotta politica e civile. La libertà è l'atmosfera nella quale le altre idee vivono e in relazione alla loro vitalità isteriliscono o si sviluppano. È l'atmosfera nella quale si vincono le battaglie dello spirito moderno».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ventesimo anniversario della morte di Giuseppe Saragat cade a pochi giorni dalla commemorazione del trentennale della morte di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta. Vorrei partire da questo strano intreccio di memoria e di ricordi, che si legano quasi in filigrana e in una sorta di sotterranea corrispondenza al sessantesimo anniversario della nostra Carta repubblicana. Dopo il settennato alla Presidenza della Repubblica, dal 1972 Saragat partecipa attivamente ai lavori del Senato, sebbene i suoi interventi acquistino il crisma dell'autorevolezza proprio perché accuratamente e ponderatamente limitati nel numero. Tra questi interventi, nel tragico 16 marzo 1978 Saragat interviene con parole vibranti per riconoscere come la strage degli uomini della scorta ed il sequestro di Aldo Moro rappresentino un «atto che colpisce al cuore il Parlamento e offende la sovranità di tutto il popolo italiano; che va combattuto con il coraggio, la forza e l'unità di tutti i veri democratici». In tale postilla si possono scorgere i tratti peculiari di tutta la sua storia e la sua biografia politica ed istituzionale. Saragat era politico, cittadino, uomo, in una straordinaria univocità di intenti, verso una proiezione ideale intrisa di valori, azione, riflessione e maturazione delle coscienze. La storia di Saragat politico si lega in modo indissolubile alla genesi ed allo sviluppo del socialismo e del Partito socialdemocratico, del quale sarà acclamato presidente il 29 luglio 1975; alla lunga sequela di incarichi di Governo degli anni Cinquanta, preceduta dall'incarico di Presidente dell'Assemblea costituente e coronata con l'elezione a Capo dello Stato del 1964; alla tenace volontà di ancorare ogni suo intervento in quest'Aula alla concretezza ed alla immediata incidenza fattuale degli avvenimenti, senza arroccarsi in peregrinazioni astratte sottratte al confronto generoso e sincero con i propri interlocutori naturali, ossia i rappresentanti dei partiti. Saragat cittadino è l'italiano combattente sull'altopiano di Asiago durante la Prima guerra mondiale; è l'italiano esiliato dal 1926, anno in cui muore Gobetti, fino al suo rientro in Italia quando viene arrestato a Susa e, dopo la lotta clandestina, di nuovo nel 1943 con Pertini, quando sarà rinchiuso nel carcere di Regina Coeli; è l'italiano liberato dai partigiani, componente del Comitato di Liberazione Nazionale, orgoglioso testimone della resistenza. Saragat uomo è l'umanista al quale Giovanni Spadolini simpaticamente rimprovera - nella pregevolissima introduzione ai discorsi pubblicati dal Senato nel 1989 la ritrosia e la timidezza a dare alle stampe le sue riflessioni maturate in esilio durante il periodo viennese, dove sotto l'influenza del socialismo austriaco anticipa gli esiti di quello che sarà definito, di lì a poco, in terra francese, 1'umanesimo marxista. Saragat uomo è l'amico di Giacomo Matteotti, Leo Valiani, Sandro Pertini. Idealmente debitore a Turati, non meno che a Croce, Einaudi e Salvemini, a Gobetti e a Gramsci, a Treves e Rosselli, Nenni, Modigliani e Buozzi. In questa vicinanza e condivisione di intenti, a tratti anche di strategie, il politico, il cittadino e l'uomo sono un tutt'uno con la storia dell'Italia, del proprio Paese che Saragat non teme di chiamare e invocare come Patria. Libertà, Patria, umanesimo, solidarietà, europeismo: lemmi di un lessico politico mai appiattito sulla contingenza, desideroso di fare del bene, fiducioso nella speranza del rinnovamento delle istituzioni. La sintesi di questo lessico civile è l'esperienza delle relazioni umane tutta interna alla dinamica politica. Contro una stereotipata e per molti aspetti convenzionale rappresentazione manichea delle contrapposizioni e della contesa dei partiti, Saragat indica una via diversa da esplorare e percorrere nella ricchezza non scontata delle sue implicazioni sul versante del governo della cosa pubblica. Questa è la via della ricerca non dei punti di frizione, ma dei punti di saldatura delle varie anime, delle diverse tradizioni, delle molte culture che modellano la vita dello Stato. Quei punti di saldatura sono la leva per il riscatto delle coscienze e la maturazione di un senso civico della comune appartenenza dei cittadini al proprio destino ed al destino della propria Patria. Destini irrinunciabilmente comuni e convergenti, che sulla scia della riflessione di Montesquieu potrebbero così sintetizzarsi: «Se sapessi di qualcosa che potesse giovare a me e riuscisse dannoso alla mia famiglia, la respingerei dalla mia anima. Se sapessi di qualcosa che giovasse alla mia famiglia non giovando invece alla mia Patria, cercherei di dimenticarla. Se sapessi di qualcosa che giovasse alla mia Patria e nuocesse all'Europa, oppure giovasse all'Europa e nuocesse al genere umano, la considererei come un delitto».

in località Mineo, provincia di Catania, in Sicilia, durante la loro attività lavorativa in una vasca di depurazione. Ricordo che il Senato ha già posto all'ordine del giorno l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle morti bianche. Invito l'Assemblea ad un minuto di silenzio in segno di cordoglio e di solidarietà nei confronti dei familiari degli operai deceduti.

sono nostri ospiti i componenti dell'Associazione Arcidonna di San Severo, in provincia di Foggia, ai quali rivolgiamo un caloroso saluto.

signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ricorre oggi il ventesimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Saragat, Presidente della Repubblica dal 1964 al 1971, uomo politico e fondatore della socialdemocrazia italiana. Figlio di immigrati sardi, proveniva da una famiglia della media borghesia italiana. Nel 1922 aderì al socialismo, non tanto per vocazione ideologica, quanto per solidarietà nei confronti della povera gente, di quel proletariato richiamato da Karl Marx che andava organizzandosi dalla fine dell'ottocento per riscattare secoli di oppressione. Socialista riformista del filone politico di Filippo Turati, divenne principale esponente del Partito socialista unitario, nato dalla scissione dei riformisti turatiani dal Partito socialista italiano, al quale apparteneva anche Giacomo Matteotti. Durante il ventennio fascista emigrò in Francia, Austria e Svizzera, stringendo con Pietro Nenni un'alleanza politica che porterà alla riunifìcazione di PSI e PSU con il Movimento di unità proletaria, dando così vita al Partito socialista

Un uomo che con scelte chiare ed inequivocabili è stato, nel corso della sua vita, sempre dalla parte giusta, a difesa della libertà politica e della giustizia sociale. Uno dei protagonisti del Novecento italiano, una figura fondamentale nella vita democratica del Paese, esecutore della maggiore evoluzione della politica in Italia nel secondo dopoguerra e nei tempi difficili della guerra fredda. Saragat è ricordato come l'artefice della svolta di palazzo Barberini, il luogo simbolo della scissione del Partito Socialista nei primi giorni del 1947, con la quale ha decretato una svolta nelle elezioni del 1948, che hanno permesso all'Italia di avere un futuro di sviluppo e di libertà nell'ambito delle democrazie occidentali. Nelle elezioni politiche del 1948 si scagliò contro il Fronte democratico popolare, l'alleanza socialcomunista in cui militava anche il "caro nemico" Pietro Nenni. Durante la campagna elettorale il Fronte gli rimproverò l'alleanza con la Democrazia cristiana, usando contro Saragat alcune espressioni denigratorie, quali socialfascista, socialtraditore, rinnegato. In quelle consultazioni il suo cartello politico, denominato per l'occasione Unità socialista, ottenne poco più del 7 per cento dei voti alla Camera dei deputati e circa il 4,1 per cento al Senato, ottenendo 43 seggi in totale nel Parlamento italiano. Riformista e dal forte senso atlantista fu favorevole al piano Marshall e all'ingresso dell'Italia nella NATO. Egli era convinto che la socialdemocrazia potesse essere politicamente un valore aggiunto e che avrebbe potuto avere una posizione elettoralmente egemonica, come del resto avveniva nei Paesi del Nord Europa. Spesso in aspra dialettica con altre forze della sinistra, egli ha tenacemente continuato nell'impegno antifascista e nel perseguimento degli obiettivi di democrazia, giustizia sociale e libertà. Più volte Vice Presidente del Consiglio nei Governi De Gasperi, fu anche Ministro degli affari esteri dal 1962 al 1964 e si schierò a favore della formula politica del centrosinistra. Il 28 dicembre 1964 fu eletto Presidente della Repubblica italiana al ventunesimo scrutinio, grazie anche ai voti decisivi dei socialisti e dei comunisti. Terminato il suo mandato nel 1971, Saragat divenne senatore a vita, ma ebbe anche l'occasione di ritornare al suo partito, di cui divenne presidente nel 1976. Non assistette alla degenerazione della politica ed alle pratiche tangentizie del cosiddetto pentapartito, decapitato a partire da 1992 dalle indagini di Mani pulite. L'attualità del pensiero e dell'esempio di Saragat rimangono con evidenza anche nell'attuale momento politico. La concretezza dell'azione, la serietà e la sobrietà del comportamento sono state l'espressione delle sue principali virtù, unanimemente riconosciute sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Anche oggi, a molti anni dalla caduta del Muro di Berlino ed all'inizio della terza Repubblica, che ha visto scomparire dalla scena politica italiana e dalle rappresentanze parlamentari non soltanto il Partito socialdemocratico, ma anche gli eredi di Filippo Turati, Pietro Nenni e Giacomo Matteotti (e non solo), occorre dare atto al pensiero di Giuseppe Saragat

fuori dalla retorica tipica di queste comemorazioni, a nostro avviso due aspetti dell'azione politica di Saragat sono particolarmente interessanti, di rilievo e di stretta attualità: il primo è l'atlantismo, la scelta occidentale che per un uomo politico di sinistra nel dopoguerra non era assolutamente scontata, anzi; il secondo è l'idea di Europa federale, l'idea di un'Europa dei popoli quale risposta al deficit democratico dello Stato nazionale.

poco importa: la storia ha dato ragione all'uomo Saragat, che non ha dovuto rinnegare imbarazzato l'appoggio all'intervento armato dei sovietici a Praga e a Budapest. Più interessante e ancora più attuale il secondo aspetto: l'idea di un'Europa federale e democratica. Saragat è nel Movimento federalista europeo, il movimento fondato da Spinelli, e con altri illustri esponenti promuove il Patto per la fondazione di uno Stato federale europeo. unico tra i 27 Paesi dell'Unione europea, si esprimerà con un referendum, democraticamente, sul Trattato di Lisbona. Questa è democrazia! Il tema del *deficit* democratico degli Stati-Nazione è quindi, cari colleghi, di stretta attualità e si lega a doppio filo con la globalizzazione. Sono democratiche le scelte prese da organismi quali il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la BCE, il WTO, il G8, la stessa Commissione europea? Nell'attuale fase postmoderna, di modernità liquida, dominata dal mito della globalizzazione, assistiamo all'inevitabile avverarsi della tesi esposta nel lontano 1995 dal grande economista Kenichi Ohmae: la fine dello Stato-Nazione e l'emergere delle economie regionali. Il sociologo Daniel Bell, americano, rileva che lo Stato-Nazione è diventato, contemporaneamente, troppo piccolo per i grandi problemi della vita e troppo grande per i piccoli problemi della vita. La sintesi l'abbiamo nell'azzeccata definizione di Robertson della "glocalizzazione", ovvero

Un esempio su tutti l'allargamento repentino a 27 Stati: va bene forse per il mercato, ma sicuramente è un freno *sine* *die* alla vera unione politica e democratica degli Stati europei. Figuriamoci se entrasse da subito la Turchia! Concordiamo quindi con Baumann: globalizzazione e territorializzazione sono due lati della stessa medaglia, due elementi dello stesso processo di redistribuzione su scala mondiale della sovranità, del potere e quindi, in ultima analisi, della libertà. Per noi della Lega Nord la strada è chiara ed è già segnata: occorre trasformare, da un lato, lo Stato-Nazione in un moderno Stato federale e, dall'altro, l'Europa delle *lobbies* e della grande burocrazia in una vera Europa federale dei popoli, politica e democratica. La storia ha dato ragione a Saragat sulla scelta atlantista. Siamo convinti che darà ragione a lui e alla Lega Nord di Umberto Bossi anche per l'idea di Europa federale dei popoli. *(Applausi

Signor Presidente, come lei ha ricordato nel suo discorso di apertura, Saragat fu il primo Presidente della Costituente. Poi ha aggiunto: Saragat, Presidente della Repubblica e, sottolineo io, primo Presidente socialista e di sinistra della Repubblica. Saragat, quindi, un socialista liberale, primo convinto sostenitore della collaborazione, per il governo del Paese, tra socialisti e cattolici democratici. Ogni volta che ci soffermiamo in una riflessione e, in un riesame del corso della vita democratica italiana dall'ultimo dopoguerra ad oggi,

Penso che sia facile, oggi, affermare che Nenni e Togliatti ebbero torto e Saragat, al contrario, fu lungimirante. se torniamo a quel momento e soprattutto al comune sentimento che la stragrande maggioranza della sinistra aveva in sé in quel tempo, constatiamo che allora

condivisa, fino ad arrivare a quella che io definisco una delle rivoluzionarie affermazioni di un altro *leader* della sinistra come fu Enrico Berlinguer,

inizialmente contrastata da gran parte della sinistra e poi condivisa, c'è stato un guardare avanti. Così pure il tema dell'Europa unita, non solo come mercato unico, ma anche e sempre più come istituzione politica;

quasi in entrambi gli schieramenti, sorge spontanea la domanda: in quale dei due campi che segnano la politica italiana oggi si collocherebbe Saragat se fosse vivo? Io non so rispondere, ma replico con una sua frase, tratta da un discorso del 1948: «Noi crediamo nella giustizia, non quella che ha la bilancia e la spada, ma quella che porta la croce di tutte le sofferenze umane, quella che ha il profumo di un pane che manca nella tavola del povero. Noi crediamo nella libertà, non quella dell'individuo chiuso nel proprio egoismo, ma quella che rileva nel volto di un proprio simile l'immagine di un volto fraterno. Noi crediamo nella pace, non in quella accidiosa dei pavidi, ma in quella dei valorosi che lottano contro il mostro della guerra per il trionfo di un mondo veramente umano». *(Applausi

a questo dibattito e che stazionano in piedi all'interno dell'emiciclo a raggiungere i propri posti o a lasciare l'Aula. Prego, senatore Vizzini. VIZZINI *(PdL)*.

mentre egli era Presidente del Partito socialista democratico italiano; partito di cui sono stato prima il vice segretario e, dopo la sua morte, ne diventai il segretario politico nazionale. Ricordo ancora la sua casa: nello studio interamente foderato di libri lungo ogni centimetro di parete, parlava senza troppe spiegazioni, segnando a dito da lontano, con singolare precisione, i volumi dai quali traeva le sue citazioni quasi tutte in lingua originale. Ho lavorato così in quegli anni con un uomo davvero particolare, che traeva la propria superiorità, che pure rischiava di dimostrarlo schivo, dal considerare la propria collocazione minoritaria nel Paese il frutto dell'illusione di una sinistra massimalista sulle masse. Indifferente a ciò, teneva ferme le proprie convinzioni ideali e si riteneva nel giusto, ostentando indifferenza, perché aveva la profonda consapevolezza che la storia gli avrebbe dato ragione. Era feroce avversario del fascismo e del comunismo, e sosteneva in ogni occasione che senza libertà e giustizia sociale non vi poteva essere democrazia. Era convinto che i socialisti democratici e riformisti avrebbero dovuto combattere insieme la propria battaglia per sconfiggere il massimalismo. In questo senso, quando ve ne furono le condizioni, incoraggiò sempre l'unità socialista, superando l'amore sviscerato e l'attaccamento alla sua creatura politica, che era il Partito socialista democratico italiano. Non fu mai un uomo che affascinò le masse, ma restò assertore convinto che alla fine i suoi avversari avrebbero riconosciuto i propri errori. Il suo sforzo era quello di mantenersi coerente e convinto di essere nel giusto: il resto sarebbe venuto poi. Tale comportamento tenne anche verso il suo partito, che fondò, guidò e tenne in vita sulla base di un carisma e una personalità che ne furono valori fondanti. Ai suoi funerali, svoltisi a piazza Navona, dopo la camera ardente allestita qui a Palazzo Madama, eravamo tutti lì, i compagni socialdemocratici che lo avevano accompagnato nel suo lungo viaggio della vita anche per brevi tratti. Neanche quel giorno a piazza Navona c'erano le masse, ci furono invece poco più di un anno dopo, in tutte le piazze del mondo democratico per salutare l'avverarsi della sua premonizione: il crollo del comunismo, simboleggiato dalla caduta del Muro di Berlino. Egli non visse abbastanza per assistervi e nei giorni della grande festa berlinese pensai a lui, mi resi conto che probabilmente Saragat quel giorno lo aveva sognato, immaginato e poi visto talmente tanto nella sua vita che non aveva neanche bisogno di assistervi davvero; lo aveva indicato con la sicurezza di sempre come ineluttabile, in ogni suo scritto, discorso e nelle dotte conversazioni con gli amici e con i compagni di partito. Forse eravamo noi e non lui ad aver bisogno di constatare che la storia gli aveva dato ragione. Saragat ha dunque assistito alla disfatta delle due più pericolose malattie del secolo scorso: il fascismo e il comunismo; da lui si deve imparare la capacità di vivere la giustezza della propria visione senza atteggiamenti di rivincita e senza nessuna forma di recriminazione. Credo che oggi qui dobbiamo ricordarlo soprattutto per i valori per i quali egli ha lottato, che sono molto di più che un partito politico e proprio per questo oggi non appartengono ad un solo partito politico: sono valori fondanti della nuova democrazia, presenti nella politica e non soltanto in una sola politica, perché il seme che Saragat ha piantato è germogliato nel grande campo di quella politica dei valori che diventa patrimonio di tutta l'umanità

Saragat, straordinario personaggio della nostra storia politica. Ricordo la sua adesione, da giovanissimo, al socialismo riformista di Giacomo Matteotti, di Turati, il suo esilio in Francia, in Austria, in Svizzera, la sua

nel lavorio diplomatico di quell'epoca per salvare Trieste e quanto fosse possibile salvare alla frontiera orientale quando sembrava che gran parte di quei territori dovesse essere occupata dalla Iugoslavia di Tito.

che sarebbe avvenuta con la cosiddetta seconda Repubblica, perché guidava un movimento politico che veniva definito "i saragattiani": nell'accezione popolare i socialdemocratici hanno coinciso, per decenni, proprio con la figura di questo grande personaggio. un uomo che anticipò, anche nella pratica, il riformismo - case, scuole, ospedali era il suo *slogan* - e non a caso si ricollegava ad una visione del socialismo, quello cui aveva aderito prima della guerra,

Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sua e dell'Assemblea su un episodio avvenuto venerdì mattina a Pagani, una cittadina in provincia di Salerno, dove un giovane ufficiale dell'Arma dei carabinieri, Marco Pittoni, che prestava il suo servizio lì solo da pochi mesi, nel tentativo di bloccare una rapina ad un ufficio postale ha affrontato, con estremo coraggio e raziocinio, e raziocinio, una banda di delinquenti, che non sono solo balordi ma hanno anche una dinastia familiare, tant'è che la persona che forse lo ha ucciso con due colpi di pistola alla gola è figlio di un *boss* della camorra di Torre Annunziata, almeno così sembra. almeno così sembra. Questo giovanissimo carabiniere, in soli pochi mesi, si era fatto rispettare dall'intera popolazione ed era conosciuto come il tenente dei bambini

pregiudicato e, dopo aver accompagnato in carcere il padre, era ritornato nell'abitazione e aveva provveduto a donare una bicicletta per cercare di far sorridere quel bambino piangente. Questo è l'ennesimo sacrificio

Qui non si trattava di un poliziotto Serpico, ma di un ufficiale dei Carabinieri che, per non creare nocumento e ulteriori problemi al pubblico e agli impiegati di quell'ufficio postale,

Credo che lei debba imporci, chiederci un minuto di raccoglimento, così come è stato fatto poc'anzi per altre ragioni altrettanto serie e invito tutti a riflettere bene sul dramma

prodigata nel manifestare ai vertici del Comando generale dei carabinieri i sensi del più profondo cordoglio e della solidarietà nei confronti dei familiari del nobile ufficiale ucciso in quello scontro.

a manifestare un momento di raccoglimento, proprio per far sentire il Parlamento sempre più vicino al dolore dei familiari e al prezzo quotidianamente pagato dalle forze dell'ordine.

L'episodio ripropone ancora una volta il triste fenomeno delle cosiddette morti bianche, sul quale lo stesso Presidente della Repubblica ha più volte attirato l'attenzione delle forze politiche e del Parlamento.

sugli infortuni sul lavoro e in particolare sulle cosiddette morti bianche. Tale proposta è stata approvata all'unanimità in tempi assolutamente rapidi, e si farà carico anche del lavoro di precedenti Commissioni istituite sullo stesso fenomeno. Mi affido, signor Presidente, alla sua sensibilità perché questa proposta possa giungere in Aula, essere discussa ed approvata nel più breve tempo possibile. Posso assicurare che da parte di tutta la Commissione che mi onoro di rappresentare c'è la disponibilità, se le norme regolamentari lo consentono, a discuterla anche immediatamente.

Presidente, per i colleghi siciliani la notizia di oggi è particolarmente grave e la ringrazio di averla ricordata all'inizio della seduta.

l'esame del provvedimento, che riteniamo assolutamente essenziale - mi rivolgo alla competenza e alla sensibilità dei colleghi della Commissione lavoro - insieme a uno studio appassionato di altre misure che possano ridurre la barbarie degli infortuni e delle morti sul lavoro.

rappresenta la prima e più urgente risposta del nuovo Governo al diffuso disagio sociale determinato dal problema della sicurezza, onorando così il prioritario impegno assunto con gli italiani. Si tratta di un disagio che nasce da problemi reali e non solamente, come spesso si afferma, da una percezione distorta di origine mediatica, come dimostrano anche recenti fatti di cronaca, che hanno visti coinvolti quali vittime perfino amministratori locali; il che, se certamente ha contribuito al successo elettorale della coalizione di centrodestra il cui approccio a tali questioni è stato evidentemente ritenuto dall'opinione pubblica più efficace e determinato - si ricollega ad esigenze che prescindono dalle divisioni di parte, tanto che non solo in buona parte il decreto-legge in conversione recepisce disposizioni che erano già contenute nel cosiddetto decreto-legge Amato, che come è noto fu emanato dal Governo Prodi e non poté essere

e ad una non aprioristica chiusura nei confronti delle nuove disposizioni e, dall'altro, una disponibilità della maggioranza a valutare positivamente le proposte del centrosinistra che risultassero migliorative del testo. Il fatto che la Commissione non abbia fatto propri gran parte degli emendamenti presentati dall'opposizione, oltre che ovviamente alla naturale dialettica fra maggioranza e minoranza e alla non coincidenza di opinioni su molte delle questioni trattate dal decreto-legge, è dipeso anche dal fatto che numerose proposte emendative del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, pur risultando dirette ad affrontare problemi cui è fortemente sensibile anche la maggioranza e spesso secondo strategie che possono apparire in gran parte condivisibili, richiedevano però approfondimenti maggiori rispetto a quelli consentiti dalla specifica sede della conversione di un provvedimento di urgenza, finendo altresì per esulare dalle materie strettamente oggetto del decreto-legge. Per quanto riguarda in particolare le competenze della Commissione giustizia, l'articolo 1 risulta composto da un unico comma suddiviso in diverse lettere, ognuna delle quali sostituisce una disposizione del codice penale. In particolare, si sono modificate le disposizioni degli articoli 235 e 312 del codice penale in materia di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero in caso di condanna alla reclusione non inferiore a dieci anni o per reato contro la personalità dello Stato. La nuova formulazione, cui la Commissione ha apportato opportuni aggiustamenti, riduce il limite di pena che consente al giudice di applicare la misura di sicurezza a due anni, introduce la previsione dell'allontanamento di cittadino appartenente all'Unione europea e aggrava la sanzione per la violazione dell'espulsione, in precedenza meramente contravvenzionale, stabilendo opportunamente la reclusione da uno a quattro anni. L'articolo reca poi una serie di disposizioni dirette ad inasprire le pene per i soggetti che abbiano commesso omicidi o lesioni colpose come conseguenza della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Va segnalato in proposito che la Commissione, approvando un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, ha elevato nel massimo la pena per l'omicidio colposo a sette anni e ciò per evitare il ripetersi di vicende, che hanno profondamente toccato l'opinione pubblica, relative all'immediata scarcerazione di soggetti che avevano commesso episodi gravi di pirateria stradale. Parimenti significative sono altre due modifiche che si propongono all'articolo 1, conseguenti rispettivamente all'approvazione di un emendamento del senatore Carofiglio e di altri senatori e di un emendamento del senatore Lumia, la prima diretta a fornire strumenti di controllo più efficaci sull'immigrazione clandestina, da un lato stabilendo adeguate sanzioni per le false o fraudolente dichiarazioni e attestazioni sulle identità proprie o di altri e, dall'altro, punendo quei comportamenti di automutilazione - in particolare, l'ustione o l'abrasione di polpastrelli - diretti a rendere più difficile l'identificazione dei soggetti. L'emendamento proposto dal senatore Lumia interviene invece sull'articolo 416-*bis* del codice penale, inasprendo le pene previste per una serie di fattispecie legate alla criminalità organizzata. La maggioranza non ha invece ritenuto di dover accogliere gli emendamenti diretti a sopprimere o modificare l'aggravante generale introdotta con la lettera *f)*, che ha istituito il numero 11-*bis* dell'articolo 61 del codice penale, prevedendo la specifica aggravante determinata dalla presenza irregolare sul territorio dello Stato, nella convinzione che tale disposizione avrà sicuramente una notevole utilità in termini di prevenzione generale. L'articolo 2 è invece intervenuto sul codice di procedura penale, da un lato estendendo il numero dei casi nei quali si procede alla distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale e dall'altra disciplinando l'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia. Anche per tale articolo, si propone una serie di miglioramenti ed integrazioni in conseguenza sia di emendamenti del Governo, sia di proposte emendative dell'Italia dei Valori. Sempre in materia di prevenzione e repressione della pirateria della strada, l'articolo 3 che sottrae al giudice di pace la competenza per le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime quando il reato sia commesso da persona che guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e l'articolo 4, che modifica in questa materia il codice della strada elevando le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Particolari problemi, onorevoli

ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; reato per cui si prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato stesso. A conclusione di un dibattito nel quale si sono manifestate numerose perplessità, sia da parte di senatori dell'opposizione che della maggioranza, sulla formulazione tecnica del nuovo reato, la Commissione ha approvato, a maggioranza, una riformulazione proposta dal Governo che, da un lato, ha chiarito che il presupposto per la verificazione del reato si rinviene nella mancanza di un idoneo titolo di soggiorno da parte dello straniero e, dall'altro, ha inserito il dolo specifico, vale a dire il fine di trarre un ingiusto profitto, così chiarendo che la norma è diretta anche a colpire lo sfruttamento delle situazioni di bisogno in cui possono versare gli immigrati clandestini. La Commissione ha inoltre approvato un emendamento proposto dalla senatrice Della Monica e da altri senatori che prende in considerazione l'ipotesi, purtroppo assai frequente, che l'immobile possa essere dato in uso ad un elevato numero di lavoratori stranieri clandestini. La Commissione ha inoltre approvato un emendamento presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori che, al fine di favorire l'identificazione e l'espulsione degli stranieri che, entrati regolarmente nel territorio dello Stato ad esempio con il visto turistico, vi si trattengono poi abusivamente, stabilendo che lo straniero proveniente da Stati per i quali è richiesto il visto d'ingresso sia sempre sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. al nostro esame reca anche importanti misure dirette a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso; in particolare, l'articolo 10 ha modificato in più punti la legge 31 maggio 1965, n. 575, per quanto riguarda le competenze delle procure distrettuali antimafia. Su tale emendamento la Commissione ha presentato una proposta di riformulazione complessiva derivante in parte da un emendamento del Governo e in parte da proposte formulate da tutti i Gruppi. Su proposta dei relatori, la Commissione ha altresì approvato un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10, al fine di rendere più efficaci le norme sulla confisca di denaro, beni ed altre utilità previste dal decreto-legge n. 306 del 1992. L'articolo 11, per il quale la Commissione, su proposta del Governo, ha approvato un emendamento che ne fornisce una formulazione più chiara, ha inteso attribuire la competenza a proporre misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 1965 ai procuratori del circondario dove dimora la persona per cui si richiede la misura di prevenzione, oltre che, beninteso, al procuratore presso il tribunale del capoluogo del distretto. L'articolo 12, infine, ha attribuito al Procuratore nazionale antimafia il potere di disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di prevenzione, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali competenti. Anche per questo articolo, la Commissione ha approvato una proposta di riformulazione presentata dal Governo. Do volentieri atto a tutti i componenti delle due Commissioni riunite 1a e 2a del massimo impegno profuso per proporre all'attenzione, alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea un testo sulla sicurezza largamente atteso dall'opinione pubblica e da tutti gli italiani. *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, il provvedimento oggetto di questa parte della mia relazione è una risposta, tempestiva quanto necessaria, che il Governo ha fornito nell'affrontare due emergenze diverse nei contenuti e nelle forme. Si tratta di fenomeni sociali che possono apparire fra loro molto distanti, ma che producono effetti che incidono drammaticamente sulla vita dei cittadini e sulla sicurezza pubblica. I lutti che flagellano, con troppa frequenza, la società interpellano la nostra coscienza di cittadini e di parlamentari e proprio per questo riteniamo nostro dovere dare risposte operative, coerentemente con il programma presentato da quella che oggi è la coalizione di Governo nel corso della recente campagna elettorale. Il primo dei temi è ben noto e riguarda l'illegalità diffusa, collegata all'immigrazione clandestina, ma anche alla criminalità organizzata, quest'ultima vero e proprio cancro della nostra società. Credo che la lotta alle mafie, comunque denominate, sia un'esigenza inderogabile di uno Stato che vuole riprendere il controllo del territorio in diverse Regioni del nostro Mezzogiorno per sconfiggere una criminalità che uccide gli uomini, ma non solo: uccide le loro libertà e quelle delle imprese, rubando il futuro alle giovani generazioni. Sono personalmente convinto che la questione delle mafie sia una ferita aperta per il buon funzionamento della nostra democrazia e che ci sia sempre più bisogno di una politica che sappia fare il proprio dovere concretamente, stando in prima linea accanto ai magistrati e alle Forze dell'ordine. Accanto a questo, vi è il tema della maggior tutela della sicurezza delle famiglie che nella loro vita quotidiana sono spesso traumaticamente sconvolte, sia nel privato delle proprie abitazioni, sia nelle strade in cui crescono incidenti di ogni tipo, con vittime sempre più numerose. Il senso di insicurezza e uno sconforto crescente della società hanno richiesto un atto immediato. Il Governo ha perciò adottato un decreto-legge per le misure più urgenti ed un disegno di legge a completamento di un intervento organico in tutta la materia. Sono convinto che debba essere apprezzata la circostanza che questo Governo, in controtendenza con un passato anche recente, ha ritenuto di dover prendere in seria considerazione idee e soluzioni efficaci proposte dall'Esecutivo precedente. Questo è il segno di una politica che ha deciso di accantonare atteggiamenti di critica pregiudiziale e che vuole misurarsi seriamente sul merito dei provvedimenti da adottare. La via intrapresa con decisione è, appunto, quella di intervenire concretamente, anche recuperando quanto di buono è stato fatto di recente. Ed in proposito voglio sottolineare come, proprio per il pacchetto sicurezza proposto dall'allora ministro dell'interno Giuliano Amato, fu imboccata all'inizio la strada del dialogo tra la maggioranza e l'opposizione di allora, ma il tentativo fu impedito dall'ostruzionismo tanto fermo, quanto cieco e sterile della sinistra massimalista. Nel riferire sui lavori delle Commissioni riunite e, specificamente, sui profili di competenza della Commissione affari costituzionali, desidero in primo luogo esprimere il mio profondo apprezzamento per il confronto pacato e fecondo tra maggioranza e opposizione su alcuni aspetti oggetto della decretazione d'urgenza. Avevamo sottolineato in Commissione, nel corso della relazione, che emergevano punti di criticità del provvedimento e di questi si è dibattuto diffusamente

ma ci siamo confrontati con grande serenità e pacatezza nel merito dei problemi. Voglio ricordare che sono stati approvati circa una quarantina di emendamenti al provvedimento e che non meno di 16 di questi sono stati presentati dall'opposizione ed approvati all'unanimità dalla Commissione su argomenti importanti come, ad esempio - ne cito uno per tutti - quello del controllo alle frontiere nell'ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari.

bene, apportando anche modifiche sostanziali all'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, potenziando gli strumenti giuridici a sua disposizione per il contrasto alla criminalità locale. Frutto di un bilanciamento tra prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e valorizzazione degli enti locali, la scelta del Governo individua nel sindaco il fulcro di una nuova sinergia nella lotta alla criminalità, soprattutto in ragione della capacità che il sindaco ha di conoscere direttamente dal territorio le problematiche che affliggono la gente. Il nuovo comma 2 dell'articolo 6, in particolare, attribuisce al sindaco il compito di concorrere ad assicurare la cooperazione tra le forze di polizia locali e statali, mentre il comma 4 amplia il suo potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, prevedendo quale situazione legittimante il provvedimento *extra ordinem* anche il pericolo grave per la sicurezza urbana. modo, l'articolo 7 attribuisce una nuova funzione ai piani coordinati di controllo del territorio, per assicurare una più intensa partecipazione della polizia municipale alle attività di tutela della sicurezza, attraverso la determinazione di rapporti di collaborazione reciproca tra la polizia municipale e la polizia di Stato. Sul tema le Commissioni riunite hanno in larga parte condiviso la *ratio* dell'intervento normativo, ritenendo però corretto accogliere una proposta di alcuni parlamentari della Lega Nord, volta a coinvolgere in quest'opera di coordinamento, oltre alla polizia municipale, anche la polizia provinciale. Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati, per cui rimando alle relazioni già svolte. Desidero anch'io sottolineare la sensibilità manifestata da tutte le forze politiche che, insieme, hanno approvato tutti gli emendamenti all'articolo 10;

gli inquirenti, la magistratura e le forze dell'ordine hanno assicurato alla giustizia i più importanti latitanti di mafia e delle altre organizzazioni di criminalità organizzata, organizzata, dando il segnale dell'inizio di una grande riscossa e rimonta sul terreno della lotta alla componente militare delle mafie, con i provvedimenti e gli emendamenti adottati all'articolo 10 si apre la caccia al tesoro delle mafie, si cerca di aprire le casseforti di Cosa nostra e delle altre organizzazioni criminali che operano sul territorio, mediante misure che possono mettere la magistratura in condizione di operare meglio, più più celermente, con minori cavilli e con grande rapidità rispetto al passato. Credo che questo sia un elemento fondamentale se si vuole puntare alla vittoria finale,

di tutti i Gruppi politici presenti nelle due Commissioni. Mi preme, peraltro, precisare che una serie di emendamenti che non hanno trovato accoglimento

nella seconda parte dell'esame del pacchetto costituito dal disegno di legge che il Governo ha già presentato e che nelle prossime settimane inizierà il suo *iter* parlamentare.

in provvedimenti specifici che potranno essere assunti. Credo che, al di là delle diversità, il dibattito nelle Commissioni riunite sia stato assolutamente positivo e che sia entrato nel merito con grande profondità.

i rappresentanti del Governo, e segnatamente i sottosegretari Mantovano e Caliendo, che non hanno mai fatto mancare in nessun minuto dello svolgimento del dibattito la loro presenza e la loro Concludo invitando l'Aula ad un dibattito sereno che non escludo potrà apportare ulteriori modifiche positive o, comunque, chiarire la portata dei problemi sui quali ci confrontiamo per dare al Paese uno strumento incisivo, moderno, che segna una nuova fase della della lotta al crimine che deve garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle famiglie per riprendere quella civile convivenza che è il punto di ripartenza di una società che vuole crescere.

per acquisire dati e notizie sul grave incidente che si è verificato in Sicilia e ha appreso che a breve il sottosegretario Viespoli, proprio a nome del Governo, si recherà

*(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico ha sollevato una questione pregiudiziale molto rilevante su questo provvedimento che riguarda il contrasto,

25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e con l'articolo 21 della Carta di Nizza. Nel merito la questione è molto semplice. La norma è con grande evidenza incostituzionale perché, sotto il profilo della determinazione della pena, prefigura una seria e infondata disparità di trattamento tra soggetti responsabili del medesimo reato; attribuisce in pratica pene diverse a seconda che si tratti di un

il Governo e la maggioranza hanno respinto in Commissione un nostro emendamento abrogativo dell'aggravante e lo hanno fatto facilmente, anche - credo - in assenza di buoni argomenti, forti della consistente maggioranza numerica. Temo

farà. In un dibattito parlamentare è fisiologico ed anche sano che maggioranza e opposizione si trovino spesso a sostenere posizioni molto lontane tra loro ed è naturale che sia così. Centrosinistra e centrodestra sono portatori di visioni politiche diverse, hanno obiettivi programmatici diversi, hanno diverse scale di priorità, ma questa legislatura è iniziata con una consistente novità, che tutti noi abbiamo rilevato con grande soddisfazione e dalla quale abbiamo ricavato speranze e aspettative per il futuro del nostro Paese: maggioranza e opposizione, e personalmente Walter Veltroni e Silvio Berlusconi, hanno annunciato la fine della stagione della contrapposizione «senza se e senza ma», della guerra ideologica e della perenne e preventiva delegittimazione dell'avversario. Ho ascoltato con attenzione il dibattito sulla fiducia e mi è sembrato molto chiaro che tutto il Parlamento abbia voluto rendere esplicito come, pur permanendo tra noi una chiara distinzione programmatica e politica, in questa legislatura prendevamo l'impegno di lavorare per riscrivere insieme le regole del gioco, senza più procedere a colpi di maggioranza. Debbo dire che per il centrosinistra questa linea è in continuità con il passato. Nella XIV legislatura - i colleghi che erano qui lo ricordano - eravamo all'opposizione ed avanzammo più volte la richiesta che sulle riforme si decidesse a larga maggioranza, ma il Governo e il centrodestra vollero modificare da soli e senza alcuno scrupolo persino larga parte della Costituzione e la stessa legge elettorale. Nella XV legislatura eravamo in maggioranza e abbiamo nuovamente chiesto la collaborazione per le riforme; non l'abbiamo ottenuta neanche quando si è trattato di correggere una legge elettorale che destra e sinistra consideravano sbagliata ed iniqua. Persino l'ultimo tentativo, quello del presidente Napolitano e del presidente Marini, è fallito per la fretta di andare alle elezioni. Adesso tutti vorremmo che questa stagione fosse terminata ed è per questo motivo che abbiamo detto basta alle contrapposizioni e all'ostruzionismo fine a se stesso. Ma ci sono alcune condizioni di sostanza fondamentali perché la nuova stagione non sia semplicemente un ennesimo evento mediatico, l'ennesimo annuncio buono solo per andare sul telegiornale delle 13 o su quello delle 20. Queste condizioni non sono nelle nostre mani di Gruppo dell'opposizione; sono tutte nelle mani della maggioranza e del Governo. La prima condizione riguarda il contenuto e la natura delle iniziative che il Governo sottoporrà al Parlamento. È necessario che non compaiano nell'ordine del giorno dei nostri lavori norme che abbiano nuovamente le caratteristiche delle leggi *ad* *personam*, che violino i princìpi del conflitto di interessi, che accentuino le disuguaglianze sociali e che, in una parola, non tengano conto dell'interesse generale del Paese. È per questo che nell'ultimo "milleproroghe" abbiamo salutato con soddisfazione il ritiro di un emendamento che prevedeva ingiusti vantaggi per il gruppo televisivo di proprietà del presidente Berlusconi. Ed è per questo stesso motivo che abbiamo denunciato - scusate l'espressione - la puzza di bruciato e l'odore nauseante degli interessi che emanava l'emendamento con il quale irritualmente, pochi giorni fa, contro la Costituzione, senza alcuna verifica tecnica preventiva, in violazione di ogni prassi e normativa amministrativa, il Governo Berlusconi, per la seconda volta in quattro anni e per motivi molto poco chiari, ha voluto regalare alla società Autostrade privilegi, vantaggi, larghi margini operativi, benefici tariffari e buoni risultati in Borsa. *(Applausi dai che può impedire il decollo della nuova stagione di rispetto e di dialogo tra centrosinistra e centrodestra. Mi riferisco alla conformità delle iniziative legislative del Governo con il dettato costituzionale, con le normative europee con i Trattati internazionali che l'Italia ha liberamente sottoscritto. Se vogliamo veramente il dialogo, se non stiamo bluffando, lo dico al Governo ed alla maggioranza, questo è un punto su cui è bene essere molto chiari. Forzature sulla costituzionalità delle leggi non solo non possono essere oggetto di trattativa, ma costituiscono una rottura, mi spiace dirlo, unilaterale di quel nuovo stile politico che tutti in teoria diciamo di volere, ma che poi dobbiamo saperci meritare con i nostri comportamenti parlamentari. Al Governo, in particolare, vorrei ricordare che su questioni delicate come quelle che riguardano la sicurezza l'Italia ha bisogno di esibire ai propri cittadini ed a tutta l'Unione europea una fedina sgombra anche del benché minimo dubbio di incostituzionalità. Norme sulle quali gravino dubbi di costituzionalità non solo corrono il rischio della censura della Corte costituzionale, ma soprattutto, e questa è, se possibile, una conseguenza ancora più grave, sono destinate a perdere il consenso dell'opinione pubblica e diventare per questo molto meno efficaci. Voglio ricordare al Ministro dell'interno (ma sono certo che lo ha ben presente) che l'Italia ha avuto negli anni Settanta il più crudele, più radicato, più diffuso terrorismo politico d'Europa. L'Italia ha battuto il terrorismo senza mai violare la sua Costituzione, senza che mai lo Stato desse la sensazione di non voler rispettare i diritti costituzionali, anche dei colpevoli, anche dei sospetti. Altre Nazioni europee sono state più disinvolte di noi, molto più disinvolte, e quei princìpi li hanno superati. Noi no, ma quella guerra l'abbiamo vinta egualmente ed oggi possiamo esserne fieri. Allo stesso modo, ne sono certo, anche la guerra alla clandestinità può essere più forte e più efficace se faremo in modo che mai nessuno possa rivolgerci l'accusa di averla combattuta in violazione della Costituzione. Ci sono quindi motivi giuridici, motivi politici ed anche motivi strategici legati alla lotta alla clandestinità che dovrebbero indurre il Senato a votare a favore della nostra pregiudiziale. Aggiungo, signor Presidente, un'ultima considerazione di carattere più politico. Tutti in quest'Aula condividiamo sinceramente l'obiettivo della lotta alla clandestinità. Il pacchetto di norme proposto dal Governo e che stiamo esaminando è tutto diretto a reprimere il fenomeno ed a colpire con più severità i clandestini sorpresi nel territorio nazionale. Lo dico senza voler dare con ciò alcun giudizio di merito. Considerata la situazione dell'ordine pubblico, il provvedimento ha una chiara natura repressiva. Il mio augurio è che adesso il Governo comprenda quanto sarebbe necessaria, terminato questo dibattito, una sua iniziativa su scala nazionale, europea ed extraeuropea che abbia l'ambizione di prevenire con efficacia la clandestinità, non solo di reprimerla dopo che si è manifestata. Se vogliamo fare sul serio dobbiamo andare alle origini del fenomeno, non limitarci a combatterne con scarsi esiti gli effetti ultimi. Perché, signor Ministro, non possiamo illuderci, la clandestinità è una delle tante forme, sia pure illegale e malata, con cui si manifestano le immense migrazioni del nostro tempo, migrazioni di interi popoli che si spostano per cercare lavoro e cibo, per paura delle persecuzioni, per fuggire alle conseguenze dei mutamenti climatici ed anche per motivi criminali. Se vogliamo incidere sul fenomeno migratorio la repressione serve a poco, a pochissimo. Investiamo sulla prevenzione. Dedichiamo alla prevenzione le nostre migliori risorse. Vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. *(Applausi

Signor Presidente, il profilo di incostituzionalità che noi solleviamo riguarda l'articolo 1 del decreto-legge. Il suddetto articolo, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, introduce l'obbligo di espulsione o di allontanamento qualora si tratti di cittadino comunitario, ricorrendo le ipotesi di condanna per un delitto contro la personalità dello Stato o per reati a pena non inferiore a due anni di reclusione. Nonostante le nostre insistenze, il Governo, con la sua maggioranza, non ha ritenuto di inserire nella norma quanto la Corte costituzionale ha affermato anche abbastanza di recente, ossia che la possibilità di espulsione o di allontanamento è subordinata all'accertamento della pericolosità sociale. Eppure, questa stessa affermazione era ed è contenuta nella relazione del disegno di legge, ove è scritto «in tutti i casi di espulsione è ormai necessario il previo accertamento giudiziale (...) della pericolosità sociale del condannato».

Io penso che la maggioranza ed il Governo lo abbiano fatto deliberatamente, perché non possono ignorare che nel 1995 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 58, pubblicata in *Gazzetta* *Ufficiale* il 1° marzo 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che prevedeva l'obbligatorietà dell'espulsione dello straniero condannato per reati collegati al traffico di stupefacenti in quanto nella norma non era contemplato l'accertamento della pericolosità sociale. Queste cose si sapevano, si sanno, ma nonostante le nostre sollecitazioni il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di non dover modificare la norma.

sanno benissimo che la Corte costituzionale non farà altro che quello che ha fatto pochi anni fa e che la stessa relazione dice, ossia ribadire la necessità di prevedere l'accertamento della pericolosità, perché è la Corte costituzionale che è intervenuta nella specifica materia. Questo è scritto a pagina 4 dalla relazione: il masochismo della maggioranza e del Governo è dunque incomprensibile, ma la serietà di noi legislatori ci impone di sollevare la questione di legittimità perché vogliamo fare le cose seriamente e, conoscendo

di difficile comprensione: mi riferisco all'articolo 5, che ha introdotto, sovvertendo il sistema, la confisca obbligatoria dell'immobile, anche escludendo la pericolosità intrinseca del bene. Si sa benissimo che la confisca è obbligatoria soltanto qualora il bene sia intrinsecamente pericoloso. Il testo proposto esclude la pericolosità del bene, però obbliga la confisca obbligatoria qualora qualcuno, come ad esempio un'anziana signora, abbia dato alloggio sotto forma di parziale retribuzione alla propria badante irregolare. Ella si vedrà condannata e vedrà il proprio appartamento confiscato. Questo avete fatto! Avete così introdotto, sovvertendo un sistema, un'ipotesi di confisca obbligatoria non prevista dalla legge e collegata esclusivamente alla nazionalità del soggetto destinatario e beneficiario del godimento dell'immobile concesso da terzi. In questo modo avete introdotto una disparità di trattamento nella qualificazione dei beni attingibili da provvedimenti ablativi della proprietà, non in virtù della qualità assegnata al bene bensì della condizione soggettiva del beneficiario e dell'utilizzazione del bene stesso. Questa è una norma profondamente incostituzionale, oltre ad essere palesemente irragionevole.

dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame del disegno di legge di conversione in quanto afflitto da pesante incostituzionalità. apre una nuova finestra"). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

pregiudiziali avanzate dai colleghi del centrosinistra, basate sulla valutazione di una presunta illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, di altre disposizioni di Trattati internazionali in particolar modo, della circostanza aggravante comune della clandestinità introdotta dal decreto-legge al nostro esame. Preliminarmente, sentiamo la necessità di ricordare che i firmatari di queste pregiudiziali di incostituzionalità

però, i loro - i vostri - decreti-legge non furono convertiti, dando un'immagine pessima del nostro Paese, un Paese che non riusciva, pur a fronte di gravissimi eventi criminosi, ad inasprire le regole di ingresso e di soggiorno degli stranieri neocomunitari. Il primo decreto-legge del Governo Prodi del 1° novembre 2007, adottato dopo il brutale omicidio a Roma di una signora italiana ad opera di un rom neocomunitario, non fu convertito. Il secondo decreto-legge del 29 dicembre 2007, adottato per rimediare alla figuraccia della mancata conversione del primo decreto-legge, non fu convertito anch'esso perché reiterare un decreto‑legge non convertito, come fece il Governo Prodi, fu davvero - quello sì - un atto costituzionalmente illegittimo. Oggi non possiamo accettare lezioni di costituzionalità sulle norme del nostro decreto-legge da parte di chi, nel 2007, non ebbe la volontà politica di affrontare il tema urgente della sicurezza, adottando un secondo decreto-legge palesemente illegittimo dal punto di vista costituzionale. I senatori Zanda, Finocchiaro ed altri sostengono che l'aggravante della clandestinità sia illegittima dal punto di vista costituzionale e che potrebbe essere legittima solo se il clandestino che commette il reato si fosse preventivamente sottratto ad un provvedimento di espulsione. Per i senatori Zanda, Finocchiaro ed altri solo in tal caso la pericolosità del clandestino sarebbe acclarata, desumendosi (riporto testualmente il periodo della vostra istanza) "da un più intenso grado di ribellione nell'azione di colui che non si è sottomesso al potere coercitivo dello Stato". Ma, colleghi, il clandestino che entra nel territorio del nostro Stato, senza alcun rispetto delle procedure, delle norme d'ingresso e di soggiorno nel nostro Stato, violando il patto di ospitalità che lo Stato ha fatto con gli stranieri con la legge Bossi-Fini (entri regolarmente se hai un lavoro, una casa e non sei un onere eccessivo per le già esigue finanze statali e comunali), il clandestino che non rispetta le nostre frontiere manifesta o no una ribellione al potere principale di uno Stato democratico, che è quello di far rispettare le proprie frontiere e quindi la sovranità dello Stato, il primo bene costituzionalmente rilevante? Ecco perché l'aggravante della clandestinità, ricollegandosi ad una condizione soggettiva di ribellione alle regole essenziali di un Stato democratico, di ribellione alla sovranità dello Stato, è legittima dal punto di vista costituzionale e per tale motivo esprimeremo un voto convintamente contrario alle questioni pregiudiziali da voi proposte. Colleghi, l'esigenza di garantire la sicurezza alle nostre famiglie assunto i caratteri della straordinaria necessità ed urgenza che legittimano pienamente il ricorso alla decretazione d'urgenza anche e soprattutto per la totale incapacità del centrosinistra nella scorsa legislatura di dare risposta al problema dell'immigrazione illegale e della criminalità organizzata di matrice straniera, indissolubilmente legata all'immigrazione illegale, come ha confermato il prefetto Manganelli nell'audizione in Commissione. L'urgenza del provvedere è quindi legata al vuoto che ci ha lasciato il Governo Prodi in tema di sicurezza; l'aggravante da applicare ai reati commessi dai clandestini è quindi una risposta dovuta al Paese e alle nostre famiglie. Chi non rispetta le nostre frontiere, chi non rispetta le nostre regole d'ingresso e di soggiorno, chi, in virtù della sua condizione di clandestinità, mette a rischio la sicurezza pubblica, manifestando un forte grado di ribellione alle nostre regole, in caso di commissione di un reato deve avere un aggravamento di pena:

Signor Presidente, signori del Governo, signore e signori del Senato, dell'intervento del senatore Zanda io ricordo poco, perché ha dedicato 45 secondi all'illustrazione della questione pregiudiziale e nove minuti e 15 secondi ad una prolusione politica che ha ricordato i loro pregi e i nostri grandi difetti. Tant'è! Per quanto attiene alla pregiudiziale che si riferisce all'aggravante, oltre a quello che ha detto il collega che mi ha preceduto, devo far notare una semplice cosa: secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, bisogna procedere, per la valutazione dell'incostituzionalità di una norma, ad una valutazione complessiva, cioè quella *secundum Constitutionem*, che è un insegnamento costante della Consulta. Ebbene, quando un soggetto si trova illegittimamente nel territorio dello Stato, significa che ha violato una legge dello Stato. Non solo, ma per valutare l'impossibile incostituzionalità dell'aggravante non possiamo dimenticare qual è la disciplina dell'articolo 59, secondo comma, del nostro codice penale, a tenore del quale delle circostanze aggravanti si risponde soltanto se se ne è a conoscenza o se si sono ignorate per colpa, il che dà

il *tertium* non è in riferimento al soggetto qualsiasi, ma al soggetto che versa *in re illicita*. Per quanto invece riguarda la questione pregiudiziale QP2, che è stata avanzata dal senatore Li Gotti e da altri senatori, sono molto perplesso e tenterò di usare la maggior cautela possibile nel ricordare che, essendo la norma sull'allontanamento del cittadino comunitario dallo Stato una misura di sicurezza, è almeno da vent'anni, dal 1986, che tutte le misure di sicurezza hanno necessariamente un accertamento di pericolosità in concreto, perché il secondo comma dell'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, ha abrogato espressamente l'articolo 240 del codice penale sulla presunzione di pericolosità. Allora, non si dica che noi vogliamo introdurre un caso di pericolosità presunta, perché non è affatto vero: proprio l'aver nominato l'allontanamento come misura di sicurezza toglie ogni perplessità al giudizio di incostituzionalità che è stato avanzato dall'Italia dei Valori, salvo errori ed omissioni (ma credo di non averli fatti). Parimenti, per quanto riguarda la confisca, l'eccezione di incostituzionalità fa riferimento più all'articolo 240 del codice penale che a dei referenti costituzionali. evidentemente il senatore Li Gotti dimentica che proprio in sede di Commissione si è provveduto, da parte del Governo, ad un emendamento che ha inserito il dolo specifico. Ed allora il bene viene adoperato al fine di un ingiusto profitto. È questo il legame che consente la confisca, perché non è più una situazione staccata dalla fattispecie, ma - come tutti quanti sanno - l'elemento soggettivo del dolo specifico illumina anche il dato sostanziale. Quindi, la confisca non sarebbe basata su nulla, ma su quella capacità criminale di sfruttamento di quel bene per il fine ingiusto.

ha espresso un giudizio ampiamente positivo sui primi provvedimenti varati dal Governo Berlusconi e volti a rafforzare la sicurezza di tutti gli italiani. Il Governo - fatemelo dire a gran voce - è partito col piede giusto; è un Governo che mantiene le promesse fatte in campagna elettorale. Non lo dico io, sono i dati a parlare e sono tutti - ma proprio tutti - dalla nostra parte. Sempre secondo Mannheimer, un sondaggista che con il centrodestra non è mai stato tenero, il consenso sulla rinegoziazione dei mutui sarebbe all'82

Se a ciò aggiungiamo che 25 elettori su 100 del Partito Democratico si dichiarano apertamente d'accordo col Governo, ciò significa che tutti quanti ci dobbiamo congratulare per l'eccellente lavoro svolto sinora dal Presidente Berlusconi e dal suo Governo. Ci ricordiamo invece cosa ha combinato il Governo Prodi in materia di sicurezza? Praticamente nulla. Ai nuovi colleghi ricordo un episodio: per adottare un decreto-legge sulla sicurezza (mi riferisco al decreto-legge c'è voluto il barbaro omicidio della signora Reggiani. Sino al giorno precedente, il Governo era riuscito, peraltro con enormi difficoltà, ad approvare soltanto dei disegni di legge. Poi, come tutti ricorderete, il suddetto decreto non è stato neanche convertito. Allora il Governo per cercare di rimediare alle divisioni presenti all'interno della sua maggioranza, ha adottato a fine anno un nuovo decreto-legge. Anche questa volta sappiamo tutti come è andata a finire: non sono riusciti a trasformare in legge neanche quel secondo decreto. Gli amici del Partito Democratico ci vengono ora a dire che sul tema della sicurezza sono uniti, perché non c'è più l'ala sinistra della coalizione. Forse loro dimenticano che assieme alla sinistra radicale essi governano Regioni, Province e Comuni. All'interno dello stesso Partito Democratico, su questo tema, ci sono - e ci sono state - forti divisioni.

del decreto-legge, noi della Casa delle Libertà, con alto senso di responsabilità, abbiamo votato la legge assieme all'allora maggioranza di Governo.

Chiusa questa breve parentesi, ritengo che lo strumento più efficace per affrontare l'emergenza sicurezza sia sempre costituito da una politica di prevenzione. I dati forniti dal Viminale mettono chiaramente in luce che la maggior parte dei reati contro la sicurezza pubblica viene messa a segno dagli stranieri: allora bene ha fatto il Governo Berlusconi, con il varo del decreto-legge, a facilitare le espulsioni dei cittadini comunitari (ad esempio, di molti rumeni) che da noi delinquono e mettono in pericolo i nostri cittadini. Chiediamo a questi ultimi di comportarsi in maniera civile o, se vogliono delinquere, di farlo nel loro Paese

gli stranieri devono sapere che in mancanza di certi requisiti (passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno) non possono soggiornare nel nostro Paese. E se lo fanno, devono essere,

i santuari dell'economia sommersa che sta distruggendo l'economia legale del Mezzogiorno e che sta rafforzando i poteri criminali, a tutto svantaggio della società onesta e laboriosa. Per queste ragioni, voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame.

il Partito Democratico considera il tema della sicurezza pubblica come una priorità assoluta, uno dei temi maggiormente sentiti dai cittadini, un problema dagli aspetti delicatissimi, perché coinvolge diritti fondamentali e inalienabili della persona umana. È con questa convinzione e consapevolezza che abbiamo affrontato il testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, di cui ci viene proposta la conversione in legge Fin dalla prima lettura del decreto-legge, anticipata peraltro da annunci e grida non sempre composti e conferenti da parte di importanti esponenti della maggioranza e del Governo, si è avuto modo di rilevare in maniera chiarissima il vuoto pressoché assoluto che caratterizzava le norme da adottare, tanto da far pensare e da farci dire che si trattava e si tratta di norme-manifesto, norme vuote, prive di contenuto e soprattutto inutili e inconferenti rispetto ai proclami lanciati ai quattro venti. Vuoto che raggiungeva il culmine con l'articolo 9 del decreto, che si limita tuttora soltanto a cambiare la denominazione delle strutture CPT senza specificarne né il contenuto né gli eventuali nuovi limiti; per di più con un atto, per definizione costituzionale, urgente e necessario come il decreto-legge. Inoltre, nelle nuove norme si ravvisavano seri profili e seri dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento in special modo alla previsione di una aggravante che sembrava quasi tirata fuori dal cilindro di un prestigiatore, ma soltanto per fare spettacolo, per colpire l'immaginazione di inconsapevoli cittadini da ingannare con il vuoto, da grida manzoniane, delle nuove norme proposte. Ben consci però dell'importanza eccezionale e della delicatezza della materia, come Partito Democratico abbiamo scelto di non alzare rigide barriere ostruzionistiche, di non fare barricate inutili. Abbiamo deciso di formulare precise proposte emendative, utilizzando esperienza e professionalità per suggerire ad un Governo, lui sì ideologico e "barricadero", le migliori soluzioni, anche tecniche, da adottare nella vastissima e multiforme problematica della sicurezza pubblica. Questo è lo spirito che ci ha animato nella stesura dei nostri emendamenti e durante le discussioni all'interno delle competenti Commissioni di merito; tuttavia, abbiamo trovato un blocco pressoché assoluto, soprattutto in ordine alle parti più qualificanti e pregnanti delle nostre proposte; un blocco per certi versi incomprensibile, come se le fila delle decisioni del Governo e della maggioranza venissero tenute da una volontà ferrea di gestire il problema-sicurezza come se si trattasse di un affare privato, quasi settario. blocco e di rigidità incomprensibili, specialmente perché, durante i lavori delle Commissioni, da più parti della maggioranza sono state formulate, *expressis verbis*, valutazioni decisamente positive in ordine ai principali emendamenti da noi proposti. Sempre nello spirito che ci ha animato dall'inizio di questa fase di lavori parlamentari, sottolineo dunque i punti fondamentali che volevamo e che vogliamo continuare a proporre. Mi limito ai principali, precisando fin d'ora che sono punti strettamente collegati a temi già trattati dal decreto-legge e da questo ritenuti necessari ed urgenti. Ogni giorno apprendiamo da stampa e televisioni di maltrattamenti e di atti di violenza gravi e gravissimi all'interno di nuclei familiari, ai danni soprattutto dei minori e delle donne, al Nord come al Sud del Paese. Sono atti vergognosi, inaccettabili, alle volte perfino raccapriccianti, oggetto ormai di lunghe ed infinite discussioni. Il Partito Democratico ha proposto e propone ancora oggi alcune norme specifiche, volte a tutelare donne e minori in tali situazioni, presentando soluzioni sia in via di prevenzione sia in forma repressiva. Che si tratti di una vera e propria emergenza come problema di sicurezza pubblica non è in dubbio; che sia necessario intervenire legislativamente con urgenza è altrettanto indubitabile. Come è possibile, signori del Governo e della maggioranza, risponderci che siete d'accordo con quanto denunciamo noi e che voi però ci state pensando, che state provvedendo e che tra breve interverrete? E intanto? Perché non ora, con lo strumento normativo più adeguato? Inoltre, ogni giorno apprendiamo da stampa e televisioni di traffici internazionali di esseri umani, traffici criminali, organizzati da bande di delinquenti situate sia in territorio nazionale che all'estero, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale, al lavoro nero; peraltro, tali traffici riguardano anche minorenni. Il Partito Democratico propone ancora oggi alcune norme precise e specifiche, volte a prevenire e a reprimere tale inaccettabile commercio di persone umane e a fornire l'autorità giudiziaria di strumenti d'intervento più efficaci. È indubitabile che si tratti di reati gravissimi ed è indubitabile l'urgenza. Non è accettabile che da parte di maggioranza e di Governo ci si dica che sono d'accordo con il contenuto delle nostre norme, ma che "loro" stanno vedendo e stanno provvedendo. Quando? Come? Banalizzando il tutto, magari con il cosiddetto emendamento Berselli-Vizzini sulle prostitute, definite pericolose ed allarmanti per la collettività, invece di decidere di intervenire subito, non contro il singolo, ma contro chi organizza e dirige questi criminali traffici internazionali. ogni giorno apprendiamo da stampa e televisioni di casi di gravi sfruttamenti del lavoro, di situazioni di caporalato, non solo al Sud ma anche al Nord (in Lombardia e in Veneto). Lavoratori stranieri, ma anche italiani, sono sottoposti a violenza, minacce, intimidazioni, sfruttando situazioni di evidente inferiorità o di stato di necessità, per di più con sistematica violazione delle normative di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quale motivo, signori del Governo e della maggioranza, dite che condividete il contenuto delle nostre proposte emendative e però non volete intervenire? Non ora, dite; e quando allora? Quanti altri crimini e quanti altri morti dobbiamo ancora aspettare prima che decidiate che ogni limite è stato superato e che la misura è colma? Non intendo dilungarmi oltremodo nell'elencazione dei nostri principali suggerimenti normativi, da voi totalmente rifiutati, anche perché potremo riparlarne in sede di illustrazione dei singoli emendamenti. Mi limito soltanto a fare cenno agli altri temi, tutti inerenti alla sicurezza pubblica, tutti urgenti, tutti necessari, da noi trattati in sede di Commissioni congiunte e da voi, con incomprensibile supponenza di tipo ideologico, rifiutati. Il Partito Democratico vi ha parlato di nuove norme sulla sicurezza stradale, sui testimoni di giustizia, sui mafiosi che continuano a godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato, di sfruttamento dei minori anche nell'accattonaggio, di rientro assistito. Niente! Avete fatto orecchie da mercante. Avete chiuso ogni porta, come se non vi interessasse la questione sicurezza, come se non vi interessasse affrontarla davvero, concretamente. Vi siete accontentati di norme di facciata, di norme‑manifesto. Non è questa la nostra linea; non è questo il nostro comportamento. Come Partito Democratico, continueremo a ragionare sul terreno dell'efficienza e della concretezza, contrastando i vostri atteggiamenti da campagna elettorale, che mirano soltanto all'effetto propagandistico e pubblicitario.

la bontà dei provvedimenti proposti dal Governo e su di essi ci siamo confrontati in Commissione e continueremo a farlo in questi giorni ostinatamente in Aula. Chiaramente, questo decreto-legge sconta un limite, cioè la sua parzialità.

la priorità vera su cui si misura il livello di affidabilità dello Stato e delle istituzioni è la capacità che ha lo Stato in tutta la sua articolazione di dare risposte certe ed efficaci al primo bisogno primario del cittadino, che è quello della sicurezza. La sicurezza, peraltro, è un'istanza sociale che riguarda soprattutto le fasce sociali più deboli, quelle che non hanno risorse per difendersi da sole e che quindi hanno la necessità di avere uno Stato forte ed autorevole che sia nelle condizioni di contrastare il crimine.

valutazione della pericolosità di alcune condotte. Quindi, è giusto che queste norme siano state inserite nel decreto-legge ed è giusto che il Parlamento su questo si confronti in maniera serena ed efficace.

prediamo intanto atto con soddisfazione dell'accoglimento di un nostro emendamento, che attribuisce ai sindaci poteri di segnalazione ai questori e ai prefetti in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. Credo che in tal modo si attribuisca ai sindaci una funzione

non possono essere esercitati dal sindaco in maniera scollegata rispetto ai poteri di direttiva del Ministero dell'interno. Infatti, se il sindaco si muove sulla stessa lunghezza d'onda del questore e del prefetto, diventando soggetto necessario dell'articolazione dello Stato in materia di contrasto e di tutela della sicurezza urbana, non è possibile che il prefetto e il questore esercitino questi poteri sotto la direttiva del Ministro dell'interno (che è autorità nazionale di pubblica sicurezza) e non altrettanto i sindaci, che con

ma, se del caso, chieda la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, affinché gli altri soggetti che fanno parte del Comitato, e quindi dello strumento di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, possano coordinare le loro azioni con quelle del sindaco. Su questo punto,

di un testo che sostanzialmente non consente di colpire tutte le ipotesi di sfruttamento illecito dell'immobile da parte del proprietario in danno dell'extracomunitario clandestino, peraltro un sistema in forza del quale, alla fine, il proprietario dell'immobile, o colui che ne ha la disponibilità, rischia di diventare responsabile penalmente, indipendentemente dalla circostanza *de facto* di

anche su quel testo. Nel momento in cui, ad esempio, si introduce il concetto di ingiusto profitto (un concetto che noi condividiamo e che giustifica l'applicazione della sanzione penale) non si può restringere l'ambito soggettivo ed oggettivo dell'applicazione della norma

sia necessario migliorare il testo. Abbiamo apprezzato il fatto che in Commissione sia stato approvato un nostro emendamento che ha previsto l'inasprimento delle pene per lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina da parte dei datori di lavoro. Abbiamo apprezzato, cioè, che non si sia colpito solo il proprietario Abbiamo apprezzato, cioè, che non si sia colpito solo il proprietario dell'immobile come fatto d'immagine, ma si sia intervenuti anche per stroncare il circuito criminogeno

*(PD)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori,

e dal senatore Casson. Pertanto, non ripeterò argomenti già trattati, ma mi limiterò a fare delle brevi osservazioni su quella parte del disegno di legge che riguarda la questione degli immigrati. È ovvio - lo do per scontato - che il nostro partito sia estremamente sensibile al tema della sicurezza,

problemi della sicurezza nel nostro Paese; se avesse messo mano alla revisione dei meccanismi di ingresso regolare, che oggi sono rigidissimi e quindi provocano un'alta irregolarità;

o dell'immigrato. Mi domando se si è mai pensato che nel nostro Paese ci sono 4 milioni di immigrati regolari con 1,5 milioni di famiglie e che abbassare così fortemente la soglia che permette l'allontanamento o l'espulsione fa rientrare nell'orbita delle persone vulnerabili familiari

senza constatare che il reato che ha commesso implica una vera e propria pericolosità sociale, allontanandolo da una famiglia che magari è italiana? Credo che questo sia un problema da tenere presente e che invece si rischia di non affrontare con questo tipo di normativa. Non parlo poi dell'aggravante comune legata all'essere irregolari nel nostro Paese (ripeto, irregolari e non clandestini); mi sembra che questo sia in qualche modo aberrante. Essere irregolari non è come compiere un delitto con crudeltà o con efferatezza o per motivi abietti o con abuso d'ufficio; è come dire che la povertà è un'aggravante. Penso che questo nasconda una ideologia veramente repressiva del tutto da respingere. Ricordo anche che per gran parte degli immigrati la caduta nello stato di irregolarità non è intenzionale, ma è dovuta alla perdita di un lavoro ed alla incapacità di ritrovare nei tempi giusti un altro lavoro che gli permetta di stare regolarmente nel nostro Paese. Infine, per quanto riguarda la cessione a titolo oneroso dell'abitazione, la riformulazione da parte del Governo non ci sembra sufficiente. Comunque c'è il pericolo di dare un segnale negativo a quei pochi proprietari di abitazioni che affittano ad immigrati e che si guarderanno bene dal metterle sul mercato bene dal metterle sul mercato per evitare ogni possibile problema con la giustizia. Credo che questo aspetto vada valutato perché potrebbe avere delle conseguenze, magari non previste ma fortemente negative.

dico anche con lealtà, comprendendo tuttavia che la situazione non è certamente uguale in tutte le parti d'Italia e dunque credo che si debbano

(al di là dell'indubbia necessità di espellere i cittadini extracomunitari clandestini che delinquono), comporta però una totale equiparazione tra questi ed i cittadini europei, al punto che un cittadino comunitario punito con una pena detentiva superiore a due anni, pur potendo non aver commesso un reato che abbia concretamente messo in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, è allontanato con un provvedimento automatico e di espulsione e con conseguente divieto di reingresso.

e recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sulla base dei quali il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato e motivi imperativi di pubblica sicurezza. Questi motivi sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero alla incolumità pubblica, rendendosi urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si tratta, quindi, di provvedimenti da motivare caso per caso da parte dell'autorità amministrativa e da valutare dall'autorità giudiziaria, come previsto dalla lettera del citato articolo 1 del decreto legislativo n. si deve tener conto dei comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino appunto una minaccia concreta ed attuale all'ordine pubblico. Vorrei ricordare che la direttiva 38 costituisce il punto di arrivo - lei lo sa benissimo, Presidente di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ai sensi della quale l'espulsione del cittadino europeo deve fondarsi su una valutazione caso per caso, di tipo soggettivo. in due sentenze della Corte di giustizia riguardanti due cittadini italiani espulsi, rispettivamente, dallo Stato tedesco e dallo Stato greco poiché avevano fatto uso di sostanze stupefacenti e commesso altri reati, sì è stabilito che, sebbene uno Stato membro possa considerare che l'uso di droghe costituisca un pericolo per la collettività idoneo a giustificare provvedimenti speciali nei confronti degli stranieri che violino la normativa sugli stupefacenti, la deroga dell'ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente. Cosicché, l'esistenza di una condanna penale può giustificare un'espulsione solo nei limiti in cui le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico.

che tutti i cittadini italiani esprimono; tuttavia, ritengo anche che si debba essere molto misurati e che il Governo, a seguito di un dibattito che mi è sembrato molto sereno - e mi auguro continui ad esserlo - voglia

queste funzionino e non siano dei meri richiami al nulla poi inapplicabili. In questo dibattito sulla sicurezza gran parte del tempo lo stiamo impegnando per parlare di immigrazione. Do per scontato che la condizione di clandestino per un immigrato non abbia e non debba avere un rilievo penale e quindi non debba essere considerata come aggravante. Cercherò di spiegare quali a mio avviso sono i punti nodali da considerare, cioè il fabbisogno dei lavoratori stranieri e la loro tutela, il continuo afflusso di stranieri clandestini e il problema della criminalità. Il nostro Paese ha bisogno di lavoratori stranieri e la domanda è sicuramente superiore al numero di ingressi regolari programmati dal Governo, tant'è che sono centinaia di migliaia gli stranieri che vivono e lavorano in Italia senza permesso di soggiorno, non per loro scelta ma per l'impossibilità di regolarizzarsi. Il meccanismo dei flussi è inadeguato e solo prevedendo un flusso continuo si abbatterebbe quasi completamente la clandestinità di chi lavora e non delinque;

da clandestini, tanto, prima o poi, ci sarà una sanatoria. Proprio questo è il punto: l'attuale legislazione favorisce l'ingresso e la permanenza nella clandestinità. Il meccanismo per cui le ambasciate italiane si dovrebbero trasformare in centri di lavoro non può funzionare, sia perché le ambasciate servono ad altro, sia perché è impensabile che un datore di lavoro per assumere un lavoratore si affidi ad occhi chiusi a chi di mestiere fa, e deve fare, altro. È ovvio, quindi, che oggi l'immigrato entri clandestinamente, acquisti fiducia presso il proprio futuro datore di lavoro spesso lavorando in nero e poi, ove riesca a superare il muro e i tempi dei flussi, si regolarizzi.

Pennapiedimonte, 600 anime, ma a forte rischio di spopolamento, il cui sindaco è andato in Romania, ha scelto dieci famiglie tra le più povere ed ora questa comunità di 45 persone vive lì, lavora e frequenta le scuole e frequenta le scuole del paese: una comunità che è considerata una ricchezza umana, sociale ed economica per quella realtà. Il sindaco di Pennapiedimonte ha potuto farlo perché i nuovi residenti sono romeni, cioè cittadini comunitari che non hanno bisogno di particolari condizioni per entrare nel nostro Paese. Ebbene, credo che vada dato più potere ai sindaci, ma ma in questa direzione, non certo per trasformarli in sceriffi. Quando uno Stato non interviene disciplinando e amministrando quelli che sono fenomeni sociali e non emergenze limitate nel tempo e nello spazio, si crea una situazione caotica in cui vige la legge del più forte: invece dello Stato di diritto si applica la legge della giungla; e chi può trarre profitto da tutto ciò se non la criminalità? Non a caso in questo nostro dibattito si è inserito il tema della prostituzione.

per prevedere che la prostituzione, quella volontaria, sia da considerarsi una professione e quindi con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono, compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale ed alla tassazione. Dobbiamo agire con la convinzione che governare i fenomeni sociali è più efficace che proibirli, nell'interesse non solo delle persone che esercitano la prostituzione o ne fruiscono, ma della società intera. Se nella clandestinità tutto è possibile, anche essere schiavi, nella legalità, con diritti e doveri, la persona è invece libera di scegliere.

voglio fin da subito esprimere il mio più vivo ringraziamento per questo provvedimento perché da tempo, da troppo tempo, il nostro Paese aspettava con ansia un'iniziativa, un provvedimento di tale portata che possa garantire la sicurezza delle nostre famiglie e di tutti i cittadini. L'apertura indiscriminata delle frontiere, il Trattato di Schengen, la globalizzazione, hanno fatto sì che nel nostro Paese sia in atto una specie di invasione di cittadini extra e neocomunitari.

e soprattutto di integrare persone che vengono da altri Paesi, con culture e tradizioni che niente hanno a che vedere con la nostra, a volte attirati dal miraggio che nel nostro Paese esista quello che alcuni definiscono il giardino dell'Eden, che si possa cioè raggiungere il benessere senza dover lavorare e produrre reddito con il sudore della fronte. Non dobbiamo farci prendere da facili sentimenti di buonismo esasperato, a volte, anzi spesso, sospinti da talune organizzazioni umanitarie che distolgono la nostra attenzione e ci fanno dimenticare che nel nostro Paese ci sono pensionati e anziani che pur avendo lavorato una vita, e taluni anche combattuto per il nostro Paese (purtroppo sono rimasti in pochi), oggi percepiscono una pensione miserevole. Invece, sempre più spesso grazie ai ricongiungimenti familiari cittadini extra comunitari, pur senza aver lavorato e versato contributi nel nostro Paese, percepiscono pensioni sociali dignitose. Signor Presidente, plaudo, anche dalla mia posizione di sindaco, alla particolare attenzione che il provvedimento in esame ha riservato agli amministratori locali, aumentando i poteri di controllo del nostro territorio.

assieme ai nostri cittadini, segnalando tutte quelle situazioni che possono essere ritenute pericolose. Ottima e sinergica è anche l'intenzione del Governo di escludere dal patto di stabilità le spese che i Comuni sosterranno per affrontare le emergenze legate ai fenomeni criminosi dei nostri paesi e delle nostre città. Non possiamo certamente avere vincoli economici quando si tratta di difendere l'incolumità dei nostri cittadini. Utilissima a tal fine è la norma del decreto che sanziona penalmente chi, dando un alloggio ai clandestini, ne favorisce la permanenza illegale nel territorio e ne approfitta dal punto di vista economico, fino ad inflazionare e a volte gonfiare il mercato immobiliare, generando fenomeni di tensione sociale laddove l'esagerata concentrazione in alloggi a volte fatiscenti innesca facilmente problemi di convivenza e spesso di tensione sociale.

che spesso e volentieri hanno provocato gravi incidenti stradali quasi sempre con il coinvolgimento di cittadini e persone estranee. Concludo dicendo che per questo, e per tanti altri motivi che verranno illustrati dai miei colleghi nel corso della discussione generale, dichiaro la piena soddisfazione del nostro Gruppo, ringraziando il ministro Maroni e tutto il Governo che ha lavorato per questo tipo di provvedimento.

provvedimenti che, causa l'interruzione anticipata della legislatura, non è stato possibile approvare definitivamente. Gli ultimi dati dicono che nel 2007 vi sono stati in Italia 2.900.000 reati, con un aumento di circa il 5 per cento rispetto al 2006 ma con un dato positivo ed in controtendenza, che dimostra come esista una strada per combattere seriamente l'insicurezza. Nelle 14 città

Questo dovrebbe portarci ad affrontare il tema della sicurezza al di fuori della logica emergenziale al di fuori di quanto un magistrato di Bologna, in un incontro svoltosi lunedì, ha definito il "carosello giudiziario" per cui ad ogni pie' sospinto si propongono nuove norme.

relatore Vizzini, il potere di ordinanza dei sindaci, pur nell'ambito di direttive che il Ministero dell'interno può dare e che secondo me è opportuno dia,

l'idea che occorra sollecitare la pubblica opinione, preoccupata per il fatto che una parte di questi reati è compiuta da immigrati clandestini, indicando negli

con l'aggravante specifica prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge, per i reati compiuti da coloro i quali sono illegalmente sul nostro territorio, che a quel reato hanno detto i colleghi ponendo le pregiudiziali. È contraria all'articolo 3 della Costituzione italiana, è contraria a tutte le norme e ai trattati internazionali, perché a seconda della condizione soggettiva della persona si determina una diversità di trattamento. Il reato di immigrazione clandestina, qualora introdotto nel nostro Paese, obbligherebbe l'apparato giudiziario, di pubblica sicurezza e penitenziario ad essere oberato di procedimenti che avrebbero come unico scopo quello di stabilire se gli oltre 700.000 immigrati irregolari che sono in Italia sono entrati legalmente o meno.

di procedimento penale per accertare se sono entrate illegalmente nel territorio nazionale, e quegli stessi anziani e quelle famiglie potrebbero essere accusate del reato di favoreggiamento.

occorre agire su due versanti. Da un lato l'immigrazione regolare va promossa e vanno modificate quelle norme assurde della legge Bossi-Fini che il centrodestra ha voluto nel 2002 e che rendono più difficile entrare nel nostro Paese

un permesso di turismo, lo lasciano scadere e poi si trattengono per cercare lavoro. È evidente allora che occorre allungare i termini dei permessi di soggiorno per ragioni lavorative, va introdotta anche la possibilità del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro e dati pieni diritti di cittadinanza agli immigrati regolari, compreso il diritto di voto alle elezioni amministrative. Dall'altro lato, quello della repressione, occorre agire con durezza su quella fascia di immigrazione clandestina che delinque e che rifiuta di declinare le proprie generalità per sfuggire ad uno o più decreti di espulsione. Questo ci dicono le autorità di pubblica sicurezza, questo ci dice la magistratura italiana*.* A noi fa piacere (lo dico qui al collega Berselli, che è stato relatore del provvedimento) che sia stato accolto dalla maggioranza e dal Governo l'emendamento 1.19, che ha come primo firmatario il collega Carofiglio. L'emendamento comporta per tutti, italiani e stranieri, un inasprimento di pena se non viene dichiarata la propria identità con la possibilità anche dell'arresto in flagranza. Questa potrebbe essere una norma importante, capace in prospettiva anche

servono solo ad agitare un simbolo nei confronti della pubblica opinione. Esse renderanno invece più difficile affrontare seriamente la questione che a parole voi dite di voler risolvere.

Signora Presidente, signori del Governo, signore e signori senatori, il pacchetto sicurezza proposto dal Governo nasce certamente da una serie di emergenze sociali, ma esso si presenta come misura strutturale nel nostro ordinamento giuridico, atta a far fronte a mutate situazioni, come ad esempio l'ampia presenza sul territorio nazionale di cittadini ormai comunitari verso i quali è tuttora necessario elevare il grado di attenzione delle forze dell'ordine. Di qui la necessità di prevedere l'espulsione, come anche quella di dare rapidità ai processi e certezza della pena. Ritengo poi importante l'aver sottolineato le responsabilità di chi trasporta i clandestini nel nostro Paese e di chi affitta loro case o alloggi approfittando anche della situazione di illegalità in cui questi soggetti vivono. Un segnale di non di poco conto è quello relativo all'aumento della pena per l'omicidio colposo commesso in violazione delle norme della circolazione stradale e sugli infortuni del lavoro. Il superamento della legge n. 626 del 1994, avvenuto recentemente, sostituita dal decreto legislativo n. 81 del 2008, aveva lasciato aperta una finestra che così si chiude. Tutto il pacchetto di norme è volto a frenare l'immigrazione clandestina e a controllare l'acquisizione della cittadinanza con provvedimenti che vanno dalla modifica del ruolo dei centri di permanenza temporanea all'azione tesa a scongiurare i matrimoni di comodo, fino alla previsione del reato di immigrazione clandestina, che verrà introdotto nel disegno di legge insieme ad altri aspetti importanti che non sono affrontati in questo decreto. Mi riferisco, ad esempio, a quelli della prostituzione o relativi alla violenza sulle donne. alla violenza sulle donne. Quest'ultimo è un fenomeno in grande espansione - lo sappiamo - purtroppo sia all'interno che fuori della famiglia; su di esso bisognerà attentamente riflettere per giungere alla predisposizione di norme atte a prevenirlo e a reprimerlo in maniera efficace. Ed è stato giusto che in Commissione si sia deciso di rinviare la materia al disegno di legge per evitare fughe in avanti su tematiche che alla che alla fine potrebbero servire solamente a guadagnare qualche titolo sui giornali se normate velocemente e non approfondite; certamente entrerebbero a far parte di quel clima di propagandismo e di campagna elettorale a cui qualcuno dell'opposizione prima ha fatto cenno.

che il sindaco può avere nell'affrontare le problematiche che si stanno adesso verificando. La seconda consiste nell'intervento volto a diminuire le vittime di incidenti stradali cagionati dall'uso e dall'abuso di alcool e stupefacenti, specialmente tra i giovani. Certo, lo Stato agisce sul fronte delle pene anche in questo ambito, in quanto deterrenti rispetto a certi comportamenti, ma è necessaria un'azione più vasta, che il Governo vuole intraprendere, vuoi per rispondere positivamente alla domanda di valori che c'è dentro a certi comportamenti giovanili, vuoi per ricostruire quel tessuto sociale che è il vero elemento efficace e di contrasto rispetto ai comportamenti criminosi. In relazione ai nuovi poteri dei sindaci, mi sento di dire che l'apporto degli enti locali può davvero costituire un valore aggiunto e il sindaco può diventare il fulcro di tale garanzia. Il sindaco è infatti in grado, più di chiunque altro, di conoscere le problematiche sociali della sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dare luogo a problemi di ordine pubblico. altresì importante che il sindaco concorra ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale, come pure che abbia il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana. Ciò è scritto nella relazione del Governo che Collegando sindaci e prefetti si consente al rappresentate dello Stato sul territorio di intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco. È di assoluta rilevanza la disposizione che prevede il potere del prefetto di indire una conferenza con i soggetti interessati, pubblici e privati, nell'ambito territorialmente interessato nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno. L'altra parte del decreto che mi sento di mettere in rilievo prevede un autonomo stato sanzionatorio per chi, guidando sotto effetto di droga o di alcool, cagiona per colpa lesioni o morte di una o più persone. Deve far riflettere la determinazione con cui il Governo vuole perseguire tali soggetti; qualcuno ha detto con il pugno di ferro: sì, credo che questo si debba proprio fare. È un provvedimento richiesto a viva voce da tanta parte della pubblica opinione, oltre che dall'Associazione delle vittime della strada. Ci rendiamo sempre più conto di come le politiche di informazione e di prevenzione e le iniziative per tutelare specialmente i giovani da una mentalità spesso nichilista semplicemente irresponsabili) non sono state sufficienti. La svolta nelle sanzioni penali, che si uniscono alle nuove sanzioni amministrative introdotte recentemente nel codice della strada, potrebbe riportare un po' di serenità in tante famiglie e far raggiungere l'obiettivo desiderato di un'ulteriore riduzione delle vittime per incidenti stradali di almeno il 50 per cento entro dieci anni. mio intervento con la richiesta di una particolare valutazione ed attenzione verso gli apolidi, verso coloro che richiedono lo *status* di rifugiato. È evidente che tale *status*, internazionalmente riconosciuto, debba mantenere anche in Italia una differenziazione rispetto a chi entra illegalmente nel Paese. È necessario, in fase applicativa, dare istruzioni ai prefetti perché vengano assicurate a tali persone le condizioni per poter vivere dignitosamente. Voterò quindi a favore della conversione del decreto-legge con convinzione e aspetto il disegno di legge, atteso da tutti i cittadini onesti a prescindere dalla propria condizione sociale. Mi auguro che su tutto il territorio venga data pronta attuazione agli strumenti che qui vengono forniti al fine di un recupero pieno della legalità e della sicurezza. Vi ringrazio, signora Presidente e colleghi, per l'attenzione.

il mio intervento oggi vuole concentrarsi prioritariamente sul tema della sicurezza stradale. Da anni assistiamo, sbigottiti e impotenti, a una serie di incidenti stradali non dovuti alla casualità o all'imperizia, ma al

Innanzi tutto, vorrei far rilevare che in sei anni questa è la terza modifica sostanziale del codice della strada e questo sicuramente non giova alla risoluzione del problema, luogo, perché vuol dire che il legislatore fa fatica a proporre una normativa efficace; in secondo la modifica continua delle norme non agevola l'informazione e la percezione che il cittadino deve avere quando si parla di regole e di comportamenti di così grave e importante significato. Le norme, soprattutto in un settore d'interesse sociale così vasto a causa della quantità dei soggetti interessati, dovrebbero essere certe, chiare e e di facile comunicazione in modo che i cittadini siano informati su regole e pratiche in maniera efficace. In fondo, è questo il motivo per cui stiamo lavorando: convincere, anche utilizzando lo strumento più estremo come la detenzione, che la tutela della vita propria e degli altri è un valore primario da difendere, anche con norme severe. È stato scritto: «Lo strumento del decreto-legge non può risolvere tutti i problemi (...) ma viene utilizzato (...) in attesa di una più compiuta rivisitazione della normativa». Queste parole, contenute nella relazione illustrativa, riconoscono che lo strumento utilizzato non è adeguato. Difficile intervenire in una materia così complessa in tutta fretta senza quella ponderazione e quel confronto necessari ad una modifica che interessi questo settore. invece, un dibattito serio ed ampio, un confronto completo tra le parti politiche nell'ambito del quale, con onestà intellettuale e politica, si sarebbero potute evidenziare le convergenze, eliminare le forzature, mettere a punto le migliori e più condivise formulazioni normative. Ma non solo. La decretazione d'urgenza non mi sembra lo strumento migliore anche perché si stanno introducendo norme, soprattutto penali, che richiedono una ben diversa organizzazione della giustizia e dell'attività di pubblica sicurezza, un apparato tecnico e professionale che deve supportare tutte le novità che si introducono, sennò rimangono lettera morta o sortiscono effetti opposti. Si pensi solo a come verrà applicato l'istituto della prescrizione in questo caso. Già da più parti si è evidenziato come l'ampliamento delle competenze dei tribunali ordinari (e questo decreto-legge ne contiene diverse) può portare a gravi ritardi o addirittura alla paralisi di alcuni uffici che già non riescono a smaltire il carico quotidiano. Io vorrei aggiungere che le misure in materia di codice della strada non possono essere efficaci se non si pensa ad un sistema diffuso di controlli, che significa più pattuglie sulla strada, strumenti tecnici disponibili, personale adeguatamente formato.

ascolto, questo dialogo tra sordi che generalmente precede poi la fase delle fatidiche votazioni. In cinque minuti, ormai ridotti a quattro minuti e mezzo, posso soltanto dare un contributo ponendomi e rispondendo con un monosillabo a tre domande politiche. La prima: bisognava dare una risposta alla domanda imperiosa di misure urgenti che viene dall'opinione pubblica nei confronti della delinquenza e dell'immigrazione sregolata, che spesso si collega con la delinquenza italiana ed importata? La risposta è sì. rappresenta una parte della risposta; si tratta di una risposta pertinente e tutte le rilevazioni, che da questo punto di vista sono un termometro che in democrazia dovrebbe avere - ci piaccia o no - il nostro ossequio e il nostro rispetto,

Può darsi che non siano tutte facilmente applicabili e semplici da far funzionare senza una grande convergenza di volontà degli apparati, della magistratura, del ceto politico, degli amministratori. Certamente è così,

crea sconquasso, si fanno muovere i cittadini e gli operatori anziché far muovere un po' alcuni magistrati. È una norma sbagliata alla quale mi opporrò anche in Assemblea. Si umilia la stragrande maggioranza dei tribunali italiani ingolfando i pochi tribunali grandi, già ingolfati, dei capoluoghi dei distretti. Si tratta - ripeto - di una norma sbagliata che, guarda caso, ha visto il consenso sia del centrodestra che del centrosinistra, come volevasi dimostrare. Terza ed ultima domanda:

dite no a tutto: il reato di immigrazione, che pure esiste in ogni Paese, non vi va bene; l'aggravante, che pure esiste ed è oggettivamente riscontrabile in tanti altri esempi degli ordinamenti giuridici penali, non vi va bene; le espulsioni, rese più facili e comunque più rigorose anche con lo *ius* magistratuale, non vi vanno bene; i centri di raccolta o di permanenza temporanea (se non

incostituzionali tanto da aver presentato una pregiudiziale. Nella sostanza permane la vostra pregiudiziale ideologica. Non ne volete far nulla e questo ci dispiace. Abbiamo fatto e facciamo bene a dialogare e a confrontarci, ma qui c'è una profonda divisione di contenuti che è giusto venga registrata dalla gente, dal popolo italiano che si è espresso poche settimane fa. È giusto che si registri che ancora non avete recepito il segnale democratico che proviene dal popolo italiano.

Prego,

lo faremo, perché su altri temi è tollerabile che non si sia in quest'Aula, ma su questo tema (ringrazio chi c'è, quindi non mi rivolgo a chi è